Grazie

nei confronti del senatore Roberto Castelli, nella sua qualità di ministro della giustizia *pro tempore*, nonché dei signori Marco Preioni, Daniela Bianchini, Fausto De Santis, Alfonso Papa, Monica Tarchi, Settembrino Nebbioso e Alberto Uva, ciascuno *in parte *in parte qua*, per i reati di cui agli articoli 110 e 323 del codice penale (abuso d'ufficio)». La relazione è stata stampata e distribuita. La Giunta delle elezioni e delle immunità ha deliberato di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Roberto Castelli nonché degli altri coindagati. L'Assemblea delibererà separatamente su ciascuna di tali proposte di diniego. Tali proposte, in base al comma 8 dello stesso articolo 135-*bis*, s'intenderanno respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, cioè 162 voti. Come stabilito ieri all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo le votazioni avranno luogo oggi pomeriggio, inizialmente con scrutinio elettronico (dando mandato al Presidente, vista la maggioranza assoluta richiesta,

sia per quanto riguarda la mattinata, sia per quanto concerne la seduta pomeridiana. Al fine di evitare incidenti, le chiederei la cortesia di essere preciso. Le decisioni della Presidenza sono d'invertire l'ordine

significherebbe che nel pomeriggio avremmo un'Aula al completo per poter votare ambedue le questioni contemporaneamente. questa inversione non risolverebbe il nostro problema, perché alle ore 16,30 ci troveremmo in piena discussione generale e l'Aula, come lei sa, signor Presidente, non sarebbe comunque in condizioni

Lei ha riassunto correttamente le indicazioni che avevo fornito. La necessità di far concludere i lavori in 1a Commissione entro pochi minuti - per le ore 11 dovremmo essere pronti, in quanto stanno definendo gli emendamenti - mi ha portato alla proposta che ho fatto.

di Ministro della giustizia *pro tempore*, nonché nei confronti di altri indagati, tutti per ipotesi di reato di cui agli articoli 110 e 323 del codice penale (concorso in abuso d'ufficio), relativamente a due consulenze affidate alla *Global Brain & Partners* S.r.l., finalizzate alla misurazione dell'efficienza del sistema giudiziario. La Giunta ha esaminato la domanda e, nel corso delle sedute del 13 e 19 dicembre 2006, è stato ascoltato il senatore Castelli, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del nostro Regolamento. Il senatore Castelli ha evidenziato come, nel periodo in cui ha svolto le funzioni di Ministro della giustizia, si sia avvalso di diverse consulenze, anche se quelle relative alla *Global Brain* sono state probabilmente le più importanti. La scelta di ricorrere a tali consulenze si inserisce nel più ampio contesto delle iniziative assunte dal Ministero, tutte finalizzate al perseguimento di un aumento dell'efficienza del sistema giudiziario. Un intervento volto a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario presupponeva - sempre secondo le affermazioni svolte dal senatore Castelli nel corso delle sedute di audizione davanti alla Giunta - la necessità di dotarsi di strumenti di analisi che permettessero di individuare le ragioni determinanti dei diversi livelli di funzionalità degli uffici giudiziari, così da poter intervenire sui punti critici valorizzando invece le soluzioni organizzative che nella prassi garantiscono maggiore efficienza. Ecco perché - sempre secondo il senatore Castelli - occorreva affrontare il problema di una misurazione dell'efficienza degli uffici giudiziari anche con il contributo di un apporto culturale innovativo che non poteva che provenire dall'esperienza del mondo dell'impresa. Quanto poi all'individuazione della *Global Brain* quale soggetto cui affidare l'attività di consulenza, il senatore Castelli ha precisato, nel corso delle audizioni davanti alla Giunta, che egli aveva avuto modo di conoscere il signor Alberto Uva e l'attività professionale dallo stesso svolta, nonché di essere altresì venuto a conoscenza che la *Global Brain* aveva ricevuto dall'Ordine degli avvocati di Milano l'incarico di compiere uno studio volto...

alle procedure e alle modalità di impiego delle risorse umane da utilizzare. Per quanto riguarda la fase di attuazione delle convenzioni, è incontestabile che l'attività amministrativa, posta in essere con la collaborazione Grazie anche al suo apporto, un sistema informatico per la misurazione del livello di efficienza degli uffici giudiziari è già stato sperimentato presso gli uffici giudiziari di Roma e di Bologna. Sto ripetendo affermazioni contenute nel testo delle audizioni svolte dal ministro Castelli, il quale, comunque, rispetto alla valutazione finale

Brain*. La richiesta di autorizzazione a procedere avanzata a carico del senatore Castelli e degli altri coindagati ritiene che la stipula della prima convenzione sia avvenuta in violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1994. In ordine all'individuazione dei predetti riferimenti normativi, è sembrato importante alla Giunta condividere le diverse conclusioni alle quali lo stesso Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma relativamente ad un altro procedimento, conclusosi con una richiesta di archiviazione nei confronti degli allora ministri della

all'interno di quella richiesta di archiviazione, ha ritenuto che la disposizione che attribuisce al Ministro, dal punto di vista sostanziale, il potere di nominare consulenti esterni debba essere individuata

inscrive appieno nei limiti di cognizione della Giunta e ciò non perché essa debba pedissequamente ripercorrere tutte le contestazioni mosse nei confronti del senatore Castelli con i capi di imputazione prefigurati dal Collegio (benché ciò venga espressamente fatto con la relazione, alla quale, comunque, rimando i colleghi che volessero approfondire la questione), ma perché, dai fatti illustrati, è possibile apprezzare il perseguimento dell'interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo e se esso, nel bilanciamento con gli altri valori in gioco, assuma o meno carattere di preminenza. In conclusione, la Giunta ha ritenuto che, pur non potendosi escludere nello svolgimento della vicenda in esame l'esistenza di profili peraltro di carattere prevalentemente, se non esclusivamente, formale - di non conformità ai parametri normativi ai quali avrebbe dovuto uniformarsi l'azione amministrativa, sostanzialmente il conferimento degli incarichi alla *Global Brain* è avvenuto senza esorbitare dai limiti imposti dalla legislazione vigente. È poi indiscutibile, secondo la valutazione della Giunta espressa a larga maggioranza, che l'attività amministrativa in questione sia stata posta in essere in vista del perseguimento di un interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo, interesse corrispondente all'esigenza di dotare l'amministrazione della giustizia di un affidabile sistema di misurazione dell'efficienza degli uffici giudiziari. Si tratta di un interesse che corrisponde ad un'antica istanza di oggettivizzazione dei parametri di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del nostro sistema di giustizia che, purtroppo, da troppo tempo è indicato al di sotto degli *standard* europei. L'esigenza di una maggiore efficienza è stata ricordata dallo stesso Presidente della Repubblica che, durante una seduta del CSM, ha testualmente affermato: «E' mia ferma convinzione che l'efficienza e la rapidità di risposta del sistema giudiziario, oltre che addurre prestigio allo stesso ordine giudiziario e consolidare così l'autonomia ordinamentale e l'indipendenza di giudizio della magistratura, costituiscano condizione essenziale per la piena realizzazione di molti altri valori di fondamentale importanza per la democrazia e lo Stato di diritto». Sul punto rinvio alla relazione perché, come tutte le contestazioni sono state in qualche modo valutate in filigrana, analizzate e considerate, così invece rispetto a questo elemento, che pure è essenziale, vi è stata una valutazione ulteriore, che è contenuta nella relazione. La ricostruzione dei fatti operata dalla Giunta consente, quindi, di ritenere che non solo l'azione del Ministro nel caso di specie è stata diretta alla realizzazione dell'interesse pubblico relativo ad un migliore e più efficiente funzionamento degli uffici giudiziari, ma che il perseguimento di tale interesse nell'esercizio della funzione di governo, nella valutazione, come ho detto, a larga maggioranza della Giunta, riveste senz'altro carattere preminente rispetto a quelle difformità dai parametri normativi di riferimento che pure potrebbero emergere dagli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, anche se - lo ribadisco - limitatamente ad alcune soltanto delle contestazioni da quest'ultima sollevate. Non spetta né alla Giunta, né al Senato, valutare se le predette difformità integrino gli estremi della fattispecie di abuso d'ufficio o se, invece, un simile esito debba escludersi alla luce di un esame degli atti, che ha indubbiamente evidenziato come alcuni aspetti di non trascurabile rilievo - della ricostruzione operata dal Collegio per i reati ministeriali siano smentiti dalle risultanze degli stessi atti trasmessi e degli ulteriori elementi acquisiti dalla Giunta. Ciò che, nel caso di specie, spetta alla Giunta e al Senato è appunto verificare se, sulla base degli atti, la condotta degli indagati risulti finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo e se, nel caso concreto, il rilievo di tale interesse rivesta carattere preminente a fronte di eventuali deviazioni rispetto al modello legale della condotta considerata. L'esito di tale verifica non può che essere positivo e indurre a ribadire conclusivamente che nella vicenda in esame il senatore Castelli e gli altri coindagati hanno agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo e che pertanto, nei loro confronti, deve trovare applicazione l'esimente di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989. Per tutte queste ragioni, la Giunta, a larga maggioranza, propone all'Aula di negare l'autorizzazione a procedere

*(Ulivo)*. Signor Presidente del Senato, onorevoli colleghi, condivido nella sostanza e nei particolari l'intervento del relatore, senatore Manzione, aggiungerò soltanto alcune specifiche ed alcune caratterizzazioni di natura tecnico-giuridica. La norma penale che è stata contestata all'allora ministro Castelli e agli altri coindagati era una fattispecie particolare, che ha sempre creato problemi anche di interpretazione e di prospettazione nell'applicazione pratica. È una fattispecie residuale, che si presenta quando non sono contestati o non possono essere contestati altri tipi di reati. Si tratta di una norma che è stata modificata alcuni anni fa dal Parlamento, proprio nell'intenzione di creare degli aspetti più rigidi e più vincolati nell'applicazione, ritenendo queste violazioni del codice penale un po' astratte, generali e generiche. In particolare, nell'articolo 323 del codice penale è inserito un requisito, quello della intenzionalità nel recare un vantaggio a terzi o nel recare danni,

più ampia: prima la procura della Repubblica di Roma e poi il Collegio per i reati ministeriali avevano avviato tutta una serie di indagini molto articolate. Alcuni procedimenti sono stati separati alcune posizioni processuali precedenti sono già state archiviate: riguardavano una serie di ex Ministri della giustizia, la cui attività è stata posta sotto la lente di ingrandimento della procura della Repubblica di Roma. Le posizioni, in particolare, come ricordava poco fa anche il relatore Manzione, riguardavano altri ministri della giustizia come Fassino, Diliberto, lo stesso Castelli; si era giunti ad una chiusura ritenendo che non ci fossero elementi per poter procedere in altro modo. Per quanto riguarda questo procedimento, è stato invece prospettato qualcosa di più, nel senso che il Collegio per i reati ministeriali ha indicato una serie di elementi indiziari che a suo giudizio potevano presentare la possibilità di una celebrazione di un processo e quindi di un dibattimento anche pubblico. Nell'ambito dell'attività della Giunta, sono state sentite tutte le persone coinvolte in questo procedimento;

È però importante dare una valutazione completa e seria in questo ambito, proprio sul contenuto della decisione del ministro Castelli per quanto riguarda il tema su cui è intervenuto.

protetto ed anche un interesse pubblico preminente. Costituisce conferma di tutto ciò proprio l'intervento che ha effettuato in quest'Aula nel gennaio scorso il ministro Mastella, che ha affrontato tematiche analoghe; ma, ancor prima dell'attuale Ministro della giustizia, sempre lo stesso ministro Castelli e, in precedenza, lo stesso Presidente della Repubblica, nonché il Consiglio superiore della magistratura hanno portato all'attenzione della cronaca

italiano. La questione è antica, per certi versi, e riguarda i parametri di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del sistema giustizia, che purtroppo, come tutti sappiamo, da troppo tempo è indicato, rispetto agli altri Paesi europei, al di sotto di *standard* accettabili, tanto che ripetutamente ci sono state condanne ad opera della Corte sovranazionale proprio per i ritardi dovuti alla mancanza di efficienza del sistema giudiziario italiano.

tra l'altro, il tema, come dicevo poco fa, è stato riproposto dall'attuale ministro della giustizia Mastella durante la seduta del Senato del 24 gennaio 2007. Quella seduta, lo ricordiamo tutti, è stata una delle principali occasioni è stata affrontata in maniera seria da quest'Aula, perché riguardava l'enunciazione delle priorità dell'azione di Governo per la giustizia. Già nel 2002, il ministro Castelli aveva affermato: «La cultura dell'amministrazione della giustizia deve essere ispirata al criterio della rigorosa valutazione della produttività degli uffici giudiziari e dei singoli magistrati che li compongono». L'esigenza di una maggiore efficienza è stata poi ricordata dallo stesso Presidente della Repubblica, che durante una seduta del Consiglio superiore della magistratura, magistratura, ha dichiarato letteralmente: «È mia ferma convinzione che l'efficienza e la rapidità di risposta del sistema giudiziario, oltre che addurre prestigio allo stesso ordine giudiziario e consolidare così l'autonomia ordinamentale e l'indipendenza di giudizio della magistratura, costituiscano condizione essenziale

parlamentari, la grande maggioranza ha votato a favore del diniego della concessione di questa autorizzazione a procedere, anche se, per doverosa cronaca, va segnalato che sono emerse alcune posizioni differenti al momento del voto, in quanto alcuni senatori della maggioranza non hanno partecipato al voto ed in quanto è stato anche rilevato che l'interesse pubblico preminente dovrebbe essere considerato e valutato in ordine, più che a un tema generale o generico, in relazione allo specifico comportamento che viene tecnicamente contestato dal Collegio per i reati ministeriali. Signor Presidente, è noto che in una materia così delicata la scelta di ogni singolo senatore non può essere assolutamente vincolata o conculcata da alcuno o da alcunché: è una questione di libera valutazione, di scelta individuale, anche se va detto che in sede di Giunta era emersa la posizione prevalente di questo Gruppo di ritenere sussistenti i presupposti richiesti dall'articolo 9 della citata legge costituzionale n. 1 del 1989. I presupposti di questo articolo 9, al comma 3, sono relativi, come si diceva poco fa, alla valutazione della sussistenza di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Dopo quello che ho poco fa riferito in ordine alle dichiarazioni ed agli interventi dell'allora ministro Castelli sia all'interno del proprio Dicastero, sia in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario; dopo quello che è stato segnalato anche dal Presidente della Repubblica all'interno del Consiglio superiore della magistratura; dopo quello che è stato ribadito dall'attuale ministro Mastella sia in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, sia all'interno di quest'Aula, credo che sia conseguente l'indicazione formulata dal nostro Gruppo di ritenere che il comportamento dell'ex ministro Castelli sia coperto dai citati requisiti e presupposti giuridici di norma costituzionale.

Presidente, credo che il collega Casson abbia già espresso le valutazioni del Gruppo dell'Ulivo, che sono largamente ricomprese nell'ampia, documentata e puntuale relazione del collega Manzione. Abbiamo valutato che, trattandosi di materie delicate, bisogna rispettare sempre le autonome coscienze dei colleghi membri della Giunta e anche dei colleghi di Assemblea, che formano la loro volontà sulla base dell'esposizione dei fatti. Il nostro Gruppo però ha fatto una valutazione di ordine generale ritenendo che non esistono in queste circostanze le condizioni per concedere l'autorizzazione. stati molto chiari sia il relatore che il collega Casson, quindi l'orientamento del Gruppo va in questa direzione, salvando le volontà dei singoli colleghi che proprio da questo dibattito possono trarre spunti di approfondimento e maturazioni di volontà di coscienza personale. Il nostro orientamento comunque va nella direzione che ho esposto.

e ho dato parere contrario all'autorizzazione a procedere, volevo confermare la contrarietà personale e - ritengo - anche di tutto il Gruppo dell'UDC. *(FI)*. Presidente, tenuto conto della relazione del relatore, si deve prendere atto che l'esito di tale verifica non può che essere positivo e indurre a ribadire conclusivamente che, nella vicenda in esame, il senatore Castelli e gli altri coindagati hanno agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico. Per questo, a nome mio e del mio partito, dichiaro di essere d'accordo con la relazione del relatore. di voto, resta stabilito, secondo quanto già comunicato e condiviso, che, con l'apprezzamento anche del Presidente, oggi pomeriggio potremo votare nel momento giusto e opportuno su questo argomento, dopo la discussione che c'è stata.

Il relatore, senatore Vitali, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La Commissione ha esaminato puntualmente una grande quantità di emendamenti, arrivando all'approvazione di alcuni di essi, che avevano ricevuto il giudizio preventivo di proponibilità; è questa una prima questione su cui vorrei intervenire. Come è noto, il disegno di legge di cui stiamo discutendo,

visto discutere sia dai banchi dell'opposizione che da quelli della maggioranza, sia noi che gli esponenti dell'attuale opposizione,

ma non è sempre facile distinguere ciò che è proroga di termini in senso proprio da ciò che è più genericamente un riferimento temporale.

ha esercitato con rigore questo esame preliminare, tant'è vero che gran parte degli emendamenti proposti inizialmente dai colleghi sono stati dichiarati improponibili.

della rilevanza e dell'importanza del vincolo stabilito dalla Costituzione all'articolo 81, secondo cui non possono essere approvati provvedimenti privi di copertura finanziaria; siamo estremamente rispettosi del lavoro e del ruolo della Commissione bilancio, che abbiamo avuto modo in varie circostanze di apprezzare. Personalmente, ieri sera ho partecipato ai lavori della Commissione bilancio e ho potuto notare lo scrupolo e il rigore con cui la Commissione bilancio, grazie ad una grande collaborazione di tutti i senatori e le senatrici, ha svolto il suo ruolo. ruolo. Il fatto che vi sia un emendamento approvato in assenza di questo parere e contro il parere della Commissione bilancio ha esclusivamente il significato di una segnalazione al fine di trovare una soluzione supportata dal parere favorevole della stessa Commissione bilancio.

per il comma 2, relativo alla cosiddetta emergenza da fronteggiare per quanto riguarda la necessità di personale infermieristico e tecnico.

del fuoco. Vi è stata invece una discussione piuttosto accesa, che sicuramente verrà riproposta negli interventi dei colleghi soprattutto dell'opposizione, per quanto riguarda il comma 5 dell'articolo 1, in base al quale si dispone che in attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti di tale Ente restino in carica fino al 30 giugno 2007, sospendendo fino a tale data le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

L'articolo 3, comma 1, su cui ancora non vi sono state particolari discussioni, dispone la proroga del termine di entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti.

abbiamo discusso in modo approfondito dei commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 3, che si riferiscono alle indennità di espropriazione e di rinuncia per quanto riguarda gli interventi statali per l'edilizia a Napoli.

Senza particolari discussioni abbiamo esaminato il comma 4 dell'articolo 3, che si riferisce alla messa a norma delle strutture ricettive.

in relazione ad un provvedimento così importante come la revisione, il riordino, lo scioglimento di una serie di organismi e di enti che, evidentemente, non svolgono più nessuna funzione e non si giustificano più.

ritengo sia molto importante, perché in questo modo il Senato può esercitare il suo ruolo su un punto davvero determinante.

Il comma 3 dell'articolo 4, riguardante la proroga di termini relativi alle indicazioni in carattere Braille su prodotti farmaceutici ed altri prodotti, non ha sollevato particolari obiezioni da parte dei colleghi.

quale stabilisce che si proroga il termine relativo ad una serie di adempimenti in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Anche a tale posso testimoniare che non è stata svolta una grande discussione. Il comma 1 dell'articolo 6, sulla protezione dei dati personali, è stato esaminato dalla nostra Commissione. Esso riguarda la proroga di termini per l'adozione del regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 2 dell'articolo 6 è piuttosto rilevante e si riferisce agli indennizzi ai profughi dalmati ed istriani. Il comma 3 dell'articolo 6 è particolarmente importante - ne abbiamo discusso - e stabilisce la proroga dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 del termine dal quale decorre il divieto di conferimenti in discarica dei rifiuti con potere calorifero superiore ad una certa quantità. di un divieto che era stato inserito nel decreto legislativo n. 36 del 2003 con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione. Il comma 4 dell'articolo 6 - tra l'altro riformulato durante l'esame della Camera e ne abbiamo discusso - estende ai cittadini dell'Unione Europea la possibilità di di usufruire dei benefici previsti per gli stranieri vittime di violenza o grave sfruttamento dall'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni Molto discusso è stato il comma 4-*bis* dell'articolo 6, che si riferisce alla proroga al 31 dicembre 2007 del termine per il transitorio mantenimento in capo alle attuali concessionarie o aziende da esse derivate

fare in modo che si tratti dell'ultima proroga e che anche il settore del trasporto pubblico locale sia messo nella condizione di poter essere oggetto di gare per quanto riguarda la gestione del servizio. So che la Commissione bilancio ha suggerito una riformulazione per quanto riguarda il comma 5 dell'articolo 6, relativo alle risorse del Ministero del commercio internazionale, a cui ci siamo uniformati. Lo stesso discorso riguarda il comma 6 del medesimo articolo 6 - risorse dell'ENAC, l'Ente nazionale per l'aviazione civile - e anche in questo caso la Commissione bilancio ha proposto una riformulazione a cui ci siamo uniformati.

Il comma 7-*bis* dell'articolo 6 riguarda la proroga del termine di presentazione delle domande di accesso al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire. Il comma 8 dell'articolo 6, oggetto di qualche osservazione da parte della Commissione bilancio, si riferisce alle modalità di utilizzo del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica. Abbiamo avuto la richiesta di una riformulazione, sempre da parte della Commissione bilancio, del comma 8-*bis* dell'articolo 6, relativo alla restituzione dei contributi pensionistici integrativi versati dai lavoratori portuali.

relativo ai benefici in favore di enti operanti nel settore della sanità privata e in situazioni di crisi, è stato discusso senza particolari osservazioni, così come l'articolo che si riferisce alla riapertura dei termini per la concessione dei benefìci antiracket e antiusura. Signor Presidente, colleghi, questo per quanto riguarda il testo del

Naturalmente si è cercato di tenere conto anche delle segnalazioni di questioni rilevanti, provenienti da senatori appartenenti alle diverse parti politiche.

l'articolo 1, al comma 1, prevedeva una proroga di termini in ordine al tetto delle spese per il personale universitario affidato al Servizio sanitario nazionale.

È stato poi approvato in Commissione un emendamento, presentato dai colleghi Mantovano, Saporito, Bianco, Pastore, Polledri, Saro e Maffioli, che si riferisce alla proroga

Vi è poi un emendamento importante presentato da moltissimi senatori e senatrici (Benvenuto, Barbolini, Bosone, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger Perrin, Rubinato, Molinari,

del termine per il risarcimento diretto relativo a sinistri che coinvolgono le macchine agricole e che quindi si riferisce ad un settore così importante come quello dell'agricoltura. poi un emendamento molto importante, che porta solo le firme dei senatori De Petris e Rossi Fernando ma che in realtà raccoglie emendamenti presentati da senatrici e senatori appartenenti a tutti gli schieramenti politici.

All'articolo 3 vi è un altro emendamento molto importante su cui la Commissione ha discusso a lungo e con grande attenzione, arrivando ad una formulazione ritenuta soddisfacente da parte di tutti. Mi riferisco

per quanto riguarda i lavori dei concessionari delle autostrade, limitatamente alle forniture ai lavori di manutenzione delle infrastrutture. In sostanza, abbiamo introdotto un limite

di approvare un emendamento relativo ad una parte di ciò che era stato proposto. Sulla rimanente parte i colleghi proponenti si sono impegnati a presentare un ordine del giorno.

e Saro). Esso è molto importante giacché si riferisce ai crediti di imposta degli investimenti nelle aree svantaggiate. Vi è un termine per il completamento degli investimenti che viene prorogato dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008.

delle camere di commercio. Si proroga il termine per l'adeguamento ad una disposizione legislativa per la quale, purtroppo, manca ancora la circolare attuativa.

Di una certa rilevanza è l'emendamento 6.7, che è stato approvato dalla Commissione e che vale a sanare un'incongruità tecnica presente nella legge finanziaria 2007 per quanto riguarda le sanzioni per il personale ai Comuni che non hanno rispettato il patto 2006.

di un disposto già presente nella nostra legislazione, cioè quello relativo all'istituzione delle tre Province di Monza e Brianza, di Barletta-Andria-Trani un emendamento dai senatori Polledri e Galli, approvato in Commissione, che si riferisce alle proroghe a termine per quanto riguarda il conferimento delle farine di origine animale,

la Commissione bilancio ha chiesto una riformulazione, il presidente Bianco, con grande

davvero, come ci ha spiegato il presidente Bianco, in qualità di proponente dell'emendamento, non vi sono maggiori oneri e quindi si è nelle condizioni di poter garantire che l'articolo 81 della Costituzione sulla copertura di spesa, approvando questo emendamento, viene sicuramente rispettato.

è stato ritirato in Commissione con l'impegno, appunto, ad una valutazione per l'Aula; il senatore Peterlini ha sostenuto, secondo me con buone ragioni e con ottimi motivi, che si tratta di uno degli aspetti importanti importanti degli accordi tra la Repubblica italiana e le province autonome di Trento e di Bolzano, che devono essere assolutamente rispettati in rapporto alle specialità ed alle autonomie di quelle Province. Province. Ho lasciato per ultima una questione rilevantissima: abbiamo esaminato e discusso un emendamento, che è stato ritirato in Commissione per poi riproporlo all'attenzione dell'Aula, inerente al tema dei *ticket* sanitari.

ad un tema estremamente sentito dall'opinione pubblica italiana, dai cittadini italiani, cioè la possibilità di introdurre misure alternative al *ticket* obbligatoriamente posto su determinate prestazioni di carattere sanitario. Desidero infine ricordare ho assunto l'impegno con la senatrice De Petris e con gli altri colleghi presentatori di riesaminare per l'Aula un emendamento discusso anche dove il proponente era l'onorevole Boato, relativo agli animali di allevamento per le pellicce, cercando sostanzialmente di introdurre una serie di misure e di norme tendenti ad allevare questi animali nelle condizioni migliori possibili.

Presidente, il mio è un richiamo al Regolamento sull'articolo 89, e in generale sulla durata degli interventi. Ho molto apprezzato, per la verità, il tono dell'intervento del relatore, che - non accade spesso - si è soffermato su tutte le questioni che sono state poste, almeno su quelle che ha ritenuto rilevanti. Vorrei sapere se è stata prevista una durata differente del dibattito, vista la lunghezza della relazione, che è durata quaranta minuti. Vorrei capire se non c'è il contingentamento dei tempi e se invece è previsto che si possa intervenire anche in difformità da quella che mi sembrava la determinazione dei Capigruppo.

e indirettamente anche al Presidente della Commissione bilancio annunciando che in particolare - se ho capito bene - su due questioni c'era bisogno di una convocazione della Commissione bilancio perché la 1a Commissione chiedeva che, in presenza di pareri espressi dalla Commissione bilancio, la stessa potesse riconsiderarli,

l'utilizzazione costruttiva e positiva del tempo che ci separa dall'inizio delle votazioni per tenere questa eventuale riunione. Chiederei solo di conoscere se la Presidenza ritiene di attivarsi.

se non sia il caso di informare il presidente Morando di questa richiesta e se non sia il caso che la Presidenza assuma delle iniziative perché effettivamente la Commissione, salvo il merito,

Le chiederei allora - se ritiene di darmi una risposta - se accoglie questa richiesta del relatore e, a questo punto, come intende proseguire,

Se esistono pregiudiziali, riterrei di procedere con l'illustrazione delle questioni pregiudiziali e con gli eventuali interventi - se ci sono - sulle stesse in discussione o in dichiarazione di voto,

alcuni aspetti del contenuto del decreto-legge che a mio avviso ne determinano una solo parziale legittimità costituzionale e comunque mostrano la mancanza di congruità del testo normativo. Innanzitutto, il decreto-legge manca del requisito della omogeneità. Infatti, il titolo del decreto-legge, confermato anche nel testo approvato dalla Camera, ha per oggetto la «proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

oppure paradossalmente proroga termini che sono già scaduti. Credo che sia difficile fare rientrare nel concetto di proroga un differimento, una dilatazione dei termini quando il termine *ad quem*, il termine finale, è scaduto e quindi l'effetto

che si riferisce al trasporto pubblico locale (vi accennava prima anche il relatore).

entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento, quindi presumibilmente a fine febbraio-inizio marzo di quest'anno, quando il termine è scaduto il 31 dicembre 2006; anche qui, un termine defunto,

di là di qualsiasi situazione che possa rientrare nel campo delle proroghe. Ad esempio, l'articolo 68-*bis* prevede la riapertura di un termine che - udite, udite - è scaduto il 28 febbraio 1999.

la delicatezza della questione, ma certamente non riguarda proroga di termini), nonché l'articolo 33-*bis*, norma interpretativa e che nulla ha che vedere con la questione termini. È quindi un provvedimento certamente non omogeneo, sicuramente più per colpa della Camera, così ligia per altro verso - almeno a suo dire - che del Governo, che in questo caso si è attenuto abbastanza rigorosamente almeno al contenuto dell'oggetto del provvedimento.

3. Essa probabilmente dovrebbe essere nota perché modifica la situazione giuridica che si è consolidata a seguito di una normativa riguardante gli interventi per la città di Napoli che mette fuori gioco - con una norma, tra altro, che mantiene l'efficacia di certe disposizioni - i diritti di soggetti che a suo tempo avevano concordato le indennità di espropriazione per interventi pubblici del territorio, sapendo che comunque l'emanazione dei decreti di espropriazione sarebbe dovuta avvenire entro un certo termine e conseguentemente avrebbero avuto un ristoro, ancorché modesto, del diritto di proprietà che in quel momento veniva compresso. Adesso si stabilisce che le che le misure previste all'epoca in questo panorama giuridico - che avrebbe comunque visto la cessazione dell'eventuale intesa

Senatore Pastore, in riferimento al già citato, dal relatore, richiamo dell'autorevole esponente della Camera, devo dire che la Presidenza, che giudica sull'ammissibilità dei suoi emendamenti in base a un Regolamento, risponde eventualmente al Presidente della Repubblica, non certo ai richiami di pur autorevoli esponenti di una Camera, che, non a caso, è definita Camera bassa. **Saluto ad una scolaresca

di Lavello, in Basilicata, cui auguro buon lavoro.

I 108 istituti sono naturalmente il nerbo della struttura del CNR. Quali rilievi di incostituzionalità si possono fare a riguardo di questa

del disegno di legge di conversione al nostro esame: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative». Qui non si prorogano termini previsti da disposizioni legislative, ma si prorogano termini previsti da un atto di gestione del CNR.

il 20 dicembre, proprio perché non erano ancora state espletate le procedure concorsuali di nomina dei direttori, che gli stessi sarebbero rimasti in carica

impedendo un periodo di *vacatio* determinato dalla scadenza degli incarichi di direzione degli istituti del predetto ente, senza che siano state definite le procedure concorsuali»: due falsità in un'unica frase. In primo luogo, non c'è nessun periodo di *vacatio,* perché, ho detto che già il 20 dicembre, prima del 28 dicembre, data del decreto-legge, il consiglio di amministrazione del CNR aveva stabilito la proroga in questione al 30 giugno 2007. In secondo le procedure concorsuali, che sono dichiarate non definite nella motivazione, sono state invece puntualmente definite e precisate e vengono sospese. A me dispiace moltissimo che vi siano falsi in atto pubblico così patenti.

per suo conto con le disposizioni adottate dal consiglio di amministrazione. Il terzo rilievo di incostituzionalità è quello relativo all'articolo 33,

proprio per garantire la libertà di ricerca e quindi una prosecuzione dell'avanzamento delle conoscenze in nessun modo limitata. Anche a questo riguardo,

Un ulteriore profilo di incostituzionalità riguarda la forma del provvedimento in esame. Si tratta, mi dicono gli specialisti, di una legge-provvedimento, una legge-provvedimento, che deve mantenere comunque i suoi requisiti di imparzialità e di uguaglianza formale anche se si riferisce ad un caso specifico, come fa in particolare in questo caso con una disposizione relativa al CNR. Quali sono le violazioni che tale legge-provvedimento riferimento al modo con cui è formulata? Innanzi tutto, c'è una violazione dell'articolo 97 della Costituzione, che vincola il legislatore ai princìpi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione. pubblica amministrazione. C'è una violazione, perché il legislatore interviene e si esprime, con questo intervento, decisamente a favore di una delle varie parti che sono in discussione e che hanno dei diritti nello specifico argomento. Pensiamo, ad esempio, a coloro che avrebbero potuto sostituire gli attuali direttori mantenuti in carica: questi signori vengono ad avere leso un loro diritto. Viene meno, quindi, il principio di imparzialità sancito dall'articolo 97 della Costituzione. Inoltre, vi è una lesione degli articoli 24 e 113 della Costituzione perché l'aver l'aver trasformato un atto sostanzialmente amministrativo, come la disposizione del consiglio di amministrazione del CNR, in atto legislativo, sottrae le conseguenze di questo atto ai normali controlli giurisdizionali. Pensate ad una persona che ritenga di essere lesa da tale disposizione: mentre se si fosse trattato di una disposizione emanata dal consiglio di amministrazione del CNR avrebbe potuto adire

Noi voteremo contro le due pregiudiziali, esposte sia dal senatore Pastore che dal senatore Possa, per motivi molto chiari e precisi che, a mio avviso, si evincono e sono stati sostanziati dall'esame in Commissione. Con questo decreto-legge si provvede a disporre la proroga in via d'urgenza, in quanto siamo pienamente nell'ambito dell'articolo 77 della Costituzione, di numerosi termini di scadenza previsti da disposizioni legislative concernenti l'attuazione di adempimenti da parte delle amministrazioni pubbliche. Questo avviene proprio al fine di corrispondere ad esigenze sopravvenute o anche di ordine sociale ed organizzativo. Il decreto-legge di proroga dei termini previsti da alcune disposizioni legislative è un testo che normalmente quest'Assemblea continuamente

Il decreto‑legge in esame rispetta anche l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, il quale, al comma 2, impedisce che per decreto il Governo possa «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 76 della Costituzione», «provvedere nelle materie indicate all'articolo 72, quarto comma, della Costituzione», «rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere», «regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti», «ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento». Tutti questi profili, assolutamente tutti,

sono chiaramente finalizzati a consentire una concreta attuazione di adempimenti

anzi secondo il relatore la necessità, di riunirsi per rivalutare i suoi pareri su eventuali riformulazioni

la Commissione bilancio ovviamente,

il rappresentante del Ministero dell'economia, ha ipotizzato che alcuni degli emendamenti su cui stavamo per esprimere, ed abbiamo poi espresso, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, potessero subire riformulazioni, in quel caso non incontrando più le obiezioni (del Governo, ed eventualmente anche della Commissione, che invece stavamo per esprimere). Noi abbiamo considerato questo argomento ma, signor Presidente, è chiaro che possiamo esaminare dei testi quando li abbiamo in mano e quando ci sono stati presentati ufficialmente.

ma è chiaro che non possiamo prendere in considerazione riformulazioni che per ora sono meramente eventuali; se passano dallo stadio virtuale di riformulazioni eventuali allo stadio reale di riformulazioni e ci vengono inviate in Commissione le esamineremo,

abbiamo espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione perché il Governo, malgrado la nostra sollecitazione, non ha presentato su quel testo la relazione tecnica. Si tratta di un emendamento che potrebbe avere un'incidenza finanziaria rilevante, anche se, per le vie brevi, al sottoscritto e ai membri della Commissione sono stati forniti argomenti a sostegno della irrilevanza della irrilevanza dei problemi finanziari sollevati da quello stesso emendamento. Tuttavia, questa irrilevanza noi la dobbiamo e la potremo valutare quando il Governo avrà presentato una regolare relazione tecnica;

se ci manda la relazione tecnica, non abbiamo alcuna obiezione a riunirci per valutare quella proposta con il massimo di obiettività. Allo stato degli atti, signor Presidente, io ho un emendamento che, presentato esattamente negli stessi termini in occasione della legge finanziaria sul medesimo tema, è stato considerato dal sottoscritto inammissibile quando era privo di copertura finanziaria e ammesso quando la copertura è stata presentata.

differente che non avrebbe motivazione per la propria diversità rispetto a quello formulato due mesi fa. Su questo punto, che so essere di grande interesse sia per la maggioranza che per l'opposizione, non c'è - lo dico chiaramente - nessun pregiudizio, siamo costretti a fare questo mestiere: se il Governo presenta la relazione tecnica nella direzione che mi si dice potrebbe essere quella della relazione tecnica, bene; in caso contrario è inutile che io riunisca la Commissione per presentarle degli argomenti che sono esattamente identici a quelli che le abbiamo già presentato questa mattina.

purché arrivino i testi che ad oggi in Commissione non sono pervenuti. Se non arrivano testi non convocherò la Commissione, non avendo alcuna ragione per cambiare alcun parere.

*(RC-SE)*. Intervengo a nome del Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea sulla questione pregiudiziale posta da due colleghi.

legati quindi all'*iter* del disegno di legge che stiamo discutendo, al fine di condizionare i tempi della sua approvazione. Si tratta ma, mi sia concesso di dire, di breve respiro, non tanto per l'economia dei nostri lavori,

Se quindi, al di là del Regolamento, potessimo discutere anche in questa sede di una pregiudiziale che definirei «politica», cioè di come anno dopo anno il cosiddetto decreto mille proroghe viene piegato alle contingenze del momento (previsioni da rivedere, testi di legge da concordare, correzioni da portare ad una finanziaria magmatica), forse - e ribadisco forse - troveremo molto convergenze, sia nelle analisi, sia nelle proposte di una possibile riforma. La stessa differenza tra i Regolamenti delle due Camere, sottolineata e richiamata dal senatore Pastore, diverrebbe un nodo politico da sciogliere e non più, invece, la solidissima ragione costituzionale, come ha ricordato durante il suo turno di Presidenza il senatore Calderoli, che ammette e consente prassi parlamentari non uniformi, ma appunto legittime, perché permesse da un Regolamento che ha valenza costituzionale. Segnalo che per quanto concerne la sua competenza, e cioè sostanzialmente il profilo finanziario, le scelte della 5a Commissione sono state improntate, come sua consolidata abitudine e come ha anche sottolineato nell'intervento che mi ha preceduto il suo Presidente, senatore Morando, al rispetto di un rigore finanziario tutto teso a non acconsentire a proposte che non abbiano una copertura finanziaria, come si dice in termini tecnici. La 5a Commissione ha quindi sicuramente adottato criteri e prodotto scelte uniformi, tanto che che rispetto ad alcune riscritture semplicemente enunciate è stato chiesto al Governo o ai presentatori di poterle tecnicamente analizzare per procedere poi a dare un giudizio compiuto.

ed il contenuto del testo e degli emendamenti - numerosissimi, tra l'altro, e sostanzialmente travalicanti la stessa materia

appare chiaro che l'unico criterio di omogeneità richiesto dal disegno di legge in questione, e quindi da rispettare, sia quello di intervenire sui termini

possono riguardare - come abbiamo visto - il patto di stabilità e alcune condizioni per gli enti locali, possono rivedere alcune scelte già assunte. Ma da questo punto di vista - ripeto - per chi è alla sua prima

volta, anche su questi provvedimenti, maggiore chiarezza, maggiore trasparenza e maggiore attinenza alla materia.